brevemente richiamata e puntualizzata, anche alla luce di alcuni avvenimenti successivi. Ad ottobre chiedevamo, insieme agli altri firmatari dell'interpellanza, quale fosse la situazione rispetto ad una serie di finanziamenti che il polo fieristico di Bologna stava attendendo. Quest'ultimo, vale ricordarlo, è un polo di attrazione internazionale, riconosciuto nel sistema fieristico mondiale per la sua alta specializzazione e per la qualità dell'offerta delle strutture e dei servizi che è in grado di mettere a disposizione. All'epoca chiedevamo quali fossero le intenzioni del Governo circa l'emanazione degli atti concernenti l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 27

decreti attuativi. Analogamente non erano stati destinati i contributi previsti all'articolo 1, comma 942, della medesima legge finanziaria,

tutte le fiere risentono in maniera molto pesante della crisi economica e la forte concorrenza già allora esercitata, in particolare per il Nord-Italia, dal polo fieristico milanese, in questo momento sta diventando estremamente dura. In Italia abbiamo un sistema che vede un'offerta di spazi fieristici esorbitante rispetto alla domanda e questo eccesso di offerta, in una fase di contrazione economica e di riduzione pesante della domanda espositiva, risulta ancora più esasperato.

sono intervenuti recentemente (prima a dicembre e poi a febbraio) due fatti che rischiano di squilibrare ulteriormente la situazione.

sembra tendere ad un ulteriore squilibrio piuttosto che ad un riequilibrio del sistema fieristico ed all'individuazione di scelte strategiche definite. È nostro interesse, quindi, capire quali siano, in generale, in ordine agli argomenti richiamati nella interpellanza di ottobre, le intenzioni del Governo relativamente agli atti di cui era attesa l'emanazione ed in particolare, con riferimento a queste ultime scelte, quali siano e come si motivino le scelte strategiche più in generale di regolazione e di supporto al sistema fieristico.

ha istituito presso l'*ex* Ministero delle attività produttive il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, finanziato con uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, prevedendo all'articolo 1, comma 3, che i criteri di riparto delle risorse del Fondo fossero stabiliti con decreto interministeriale tra il predetto Ministero, di concerto con il Ministero dei trasporti ed infrastrutture. Detta legge aveva di fatto individuato quali destinatari di specifici interventi per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, senza stabilirne l'entità, anche le fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova. La stessa legge n. 105 del 2006 aveva poi previsto all'articolo 1, comma 3, che dalle risorse del Fondo venisse destinato alla realizzazione di infrastrutture al servizio della fiera di Bologna un importo pari a 3 milioni di euro per il triennio 2005-2007. Di queste risorse sono rimasti, come residui Per evitare di perdere la disponibilità di tale importo, il Ministero dello sviluppo economico l'ha comunque impegnato entro il termine prescritto del 31 del 31 dicembre 2008. È stata, infatti, attivata per il triennio 2005-2007 una concessione provvisoria alla Regione Emilia-Romagna per la fiera di Bologna, condizionandone l'erogazione e l'utilizzo all'approvazione dei criteri di riparto, previsti dal decreto interministeriale in questione. La legge finanziaria 2007 aveva provveduto a rifinanziare il predetto Fondo con un ulteriore stanziamento di tre milioni di euro per 15 anni, a decorrere dal 2007, nello stato di previsione di spesa del Ministero dei trasporti ed infrastrutture. Su tali risorse, in base a quanto comunicato dai rappresentanti di tale Ministero, con successivi interventi legislativi, sono stati operati tagli che di fatto hanno azzerato ogni disponibilità per gli esercizi 2009-2011. Per tale motivo, la fiera di Bologna non ha potuto beneficiare dei contributi per la realizzazione di infrastrutture. Tale situazione è emersa quando lo schema di decreto interministeriale di riparto delle risorse del Fondo è approdato al vaglio della Conferenza unificata. In tale occasione, in data 8 gennaio 2009, è stata evidenziata dal Ministero dell'economia la necessità di una rielaborazione del testo del decreto con una nuova modulazione delle risorse assegnate al Fondo. Il Ministero dello sviluppo economico ha quindi provveduto ad avviare contatti informali sia con gli uffici del Ministero dei trasporti che con le strutture del coordinamento regionale (tenuto conto della competenza regionale in materia fieristica) per pervenire ad un nuovo testo di decreto interministeriale di riparto del Fondo, sulla base delle risorse disponibili. Dette risorse sono riconducibili ai 3 milioni nella disponibilità del Ministero dello sviluppo economico ed impegnati a favore della Regione Emilia-Romagna, e ad ulteriori 3 milioni di euro, quale residuo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa 2008 del Ministero dei trasporti, non ancora impegnati. Il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre, per quanto riguarda la concessione di contributi agli enti fieristici per potenziare l'attività di promozione e di sviluppo del *made in Italy,* anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico, emanato il decreto ministeriale n. 83 del 2008 (in attuazione della legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 942), autorizzando quindi uno stanziamento nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro. Tale decreto prevede un bando di gara, al fine di stabilire i criteri di redazione dei progetti e i parametri per la formazione delle graduatorie per l'attribuzione dei relativi finanziamenti. A tale proposito, occorre segnalare che è in corso un'iniziativa di carattere normativo, attualmente all'esame del Senato nell'Atto Senato n. 1195, intesa a consentire che le risorse, pari a dieci milioni di euro, previste, come detto, dalla finanziaria del 2007 e prive di copertura, gravino sulle economie derivanti dalle revoche dei programmi agevolati ai sensi della legge n. Solo dopo la definizione di tale iniziativa normativa e la soluzione dei problemi di copertura finanziaria potrà essere effettuata l'emanazione del bando di gara previsto dal decreto ministeriale n. 83 del 2008. Il Ministero dello sviluppo economico, comunque, continuerà ad attivarsi al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per l'attuazione di tale provvedimento, tenendo in massimo conto il processo di internazionalizzazione del sistema fieristico italiano. Basta ricordare che, in attuazione dell'accordo di settore tra il Ministero, le Regioni e le Province autonome, l'Associazione esposizioni e fiere sono stati approvati, nel periodo 2005-2008, 62 progetti di fiere, volti alla promozione delle manifestazioni sui mercati esteri (con un accantonamento sul programma promozionale ICE pari a 9.500.000 euro per gli anni 2005‑2008). Si ricorda, in conclusione, che la fiera di Bologna è stata già coinvolta in 11 iniziative progettuali, collocandosi al primo posto tra i soggetti beneficiari dell'intervento, seguita dalla fiera di Parma, da quella di Rimini e da quella di Verona.

Mi pare che il quadro che viene proposto non si discosti dalla descrizione che era già contenuta nell'interpellanza. Lo stato dell'arte - purtroppo temo temo non sia un errore quanto il Sottosegretario sottolineava - è che i 3 più 3 milioni di euro, già teoricamente previsti

Sono 3 milioni di euro e sono rimasti tali perché mai nulla è stato erogato. Il saldo, cioè, è pari a tre milioni perché non sono state erogate risorse. Mi pare invece grave che *ex post* si assuma il fatto che riparti e stanziamenti, che erano già previsti, siano completamente privi di copertura; copertura che è stata trovata per altre destinazioni. Le citate citate fiere di Verona, di Padova, di Foggia e di Bari, che pure erano tra le destinatarie previste dagli interventi del

capito, dall'Atto Senato n. 1195, che peraltro contiene moltissime altre materie. Io non posso fare altro che assumere queste informazioni

coerenti con una distribuzione territoriale sensata e attenta ad ad orientare in termini produttivi e proattivi il complesso delle risorse destinate ai moltissimi poli fieristici presenti. Segnalo che sugli ultimi temi posti, e quindi sullo scoperto che riguarda le destinazioni per la fiera di Bologna, a fronte delle risorse ritrovate per gli altri poli fieristici citati, quelli veneti e quelli pugliesi, è stato presentato da altri colleghi un analogo atto di sindacato circa 20 giorni fa. Spero che il Ministero in quell'occasione, rispondendo il più celermente possibile a questa nuova richiesta di chiarimenti, possa concretamente mettere mettere in campo interventi che vadano a sanare uno squilibrio assolutamente evidente che pesa non solo sulla fiera di Bologna, ma sul complesso degli interventi a supporto dello sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna e delle aree che con la Regione Emilia Romagna scambiano. Ricordo che le fiere dell'Emilia-Romagna costituiscono uno dei portali più importanti rispetto all'oriente, inteso sia come Europa orientale che come Estremo Oriente. In questa fase di

In via preliminare, si fa presente che i commi da 143 a 149 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 prevedono una serie di meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Tali disposizioni hanno trovato attuazione nel decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio scorso e, nel decreto interministeriale, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica, recentemente firmato dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per quanto riguarda l'emanazione dei decreti attuativi di competenza primaria del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui alla legge n. 222 del 2007, la predetta amministrazione ha precisato che nel corso dell'anno 2008 ha svolto un lavoro tecnico di approfondimento interministeriale, anche con la partecipazione degli operatori interessati. In considerazione delle esigenze espresse dalle altre amministrazioni coinvolte, a fine 2008 sono state definite, quindi, proposte emendative della norma, capaci di migliorarne l'efficacia applicativa. Il citato Ministero ha, altresì, comunicato che è in via di predisposizione la bozza di decreto attuativo, diretto a dare esecutività alle disposizioni normative, relative alla promozione dell'energia elettrica da biomasse di filiera corta. Secondo quanto precisato, tale bozza, entro la fine del corrente mese di marzo, verrà diramata per la condivisione interministeriale e la successiva presentazione agli operatori interessati. Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 3 del disegno di legge, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare»,

rendendo tali incentivi immediatamente operativi per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW. Nel caso di approvazione di tale disegno, nella sua forma attuale, dunque, non sarebbe più necessaria l'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole per consentire l'accesso agli incentivi. Si fa, comunque, presente che il citato decreto attuativo del 18 dicembre 2008 prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto di competenza del Ministro delle politiche agricole, ovvero dell'approvazione del sopraccitato disegno di legge, sia riconosciuto anche alle biomasse da filiera il valore "base" degli incentivi, subordinando il riconoscimento della tariffa maggiorata all'eventuale emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole.

non risultava a quella data emanato alcun decreto ministeriale attuativo. Prendo atto che il Governo - nella fattispecie il Ministero dello sviluppo economico - ha provveduto ad emanare un primo decreto, quello citato del 18 dicembre che è condizione primaria per concretizzare i meccanismi di incentivazione previsti ed anche gli ulteriori provvedimenti che riguardano il fotovoltaico.

il Paese si è dato per l'Europa per il 2020, con incentivi che devono andare ben oltre in obiettivi e in impegno. Riteniamo che vi sia l'esigenza di rivedere

veri e propri pionieri sul territorio, utilizzando materiale che proviene dal sottoprodotto delle filiere agricole. Hanno dimostrato con grande caparbietà che è possibile ottenere uno stato di equilibrio importante nel produrre energia senza andare in concorrenza con le filiere alimentari

relativamente al servizio pubblico radiotelevisivo siano quelle previste dalla legge e dal contratto di servizio, con il quale sono individuati gli specifici diritti e obblighi della società concessionaria. Con particolare riferimento alla attività di vigilanza e controllo, il Testo unico della radiotelevisione affida alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato conformemente al dettato normativo e al contratto nazionale di servizio, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo. In base al contratto di servizio vigente, poi, il Ministero è tenuto a curare la corretta attuazione degli obblighi in esso previsto, senza tuttavia potere intervenire su aspetti che esulano dallo stesso quale deve intendersi la determinazione dei compensi artistici, rimessa alla libera scelta imprenditoriale dell'azienda e dunque dei suoi organi a ciò preposti. In merito ai compensi percepiti dal signor Paolo Bonolis per la conduzione del Festival di Sanremo, appare poi opportuno rammentare che, in piena ottemperanza alla normativa in essere, i limiti alle retribuzioni non riguardano i compensi artistici. Essi, infatti, sono ovviamente legati a regole di mercato, dettate anche dalla concorrenza. La RAI, anche in tempi di crisi, come quelli attuali, non può autonomamente sottrarsi a tali regole, pena un decadimento della qualità della produzione, che provocherebbe in termini di immagine, di *audience* e dei conseguenti mancati introiti pubblicitari, danni ben più gravi del livello del compenso riconosciuto comunque ad un artista di elevato spessore professionale e in possesso di un forte consenso popolare. In particolare, è opportuno considerare come il Festival di Sanremo rappresenti l'evento più rilevante della programmazione RAI e costituisca sia una componente dell'offerta di servizio pubblico (in quanto evento di interesse generale, da diffondere necessariamente in chiaro), sia un elemento chiave per gli introiti commerciali e pubblicitari (complessivamente quantificabili nell'ordine di circa 19 milioni di euro). Il signor Bonolis è sia conduttore che direttore artistico del Festival, oltre che artista di fama riconosciuta, e il compenso negoziato è, da un lato, inferiore ai valori di mercato e, dall'altro, pari a quello riconosciuto per l'edizione precedente. A tal proposito, si segnala che, in termini di ascolti, l'edizione 2008 ha conseguito una media di poco più di 6 milioni di 6 milioni e mezzo di spettatori, pari ad una *share* del 35 per cento, mentre quella del 2009 ha raggiunto un ascolto medio di quasi 10 milioni e mezzo di spettatori, pari al 48 per cento di *share*; l'edizione 2009, in definitiva, ha consentito di incrementare il risultato medio di ascolto di quasi 4 milioni di spettatori, corrispondenti a 13 punti percentuali di *share*. Un altro elemento importante è dato dal fatto che l'edizione 2009 ha consentito di invertire il *trend* calante degli ascolti che durava dal 2003, con la sola eccezione dell'edizione del 2005 (peraltro condotta anch'essa da Paolo Bonolis). Relativamente alla prestazione di Roberto Benigni si segnala che l'importo riconosciuto (pari a 350.000 euro) è inferiore a quello (di 450.000 euro) riconosciuto nel 2005 per la partecipazione dello stesso Benigni a «Rock Politik» e comunque fa riferimento a un artista tradizionalmente e strategicamente legato alla RAI, oltre che a uno dei massimi professionisti italiani del settore. Sotto questo profilo, ancora, si segnala che la concessionaria SIPRA ha quantificato in almeno un milione di euro il danno che la RAI avrebbe subito senza la partecipazione di Benigni a Sanremo, non considerando peraltro gli impatti di carattere più strategico che si sarebbero venuti a determinare sul tema del rilancio del Festival (obiettivo che, come visto con i risultati di ascolto sopra sintetizzati, può dirsi pienamente raggiunto). Il complessivo valore strategico dell'operazione - come detto, più volte ribadito dalle strutture editoriali e di rete - è il legame anche con il rilancio del Festival nel Comune di Sanremo (con il quale è già stato approvato dal Consiglio di amministrazione della RAI il rinnovo della convenzione triennale) e comporta vantaggi per la RAI sia in termini di immagine, sia per la raccolta pubblicitaria. Aspetto questo ultimo che non va sottovalutato in considerazione dell'attuale periodo di profonda crisi economica del Paese. In conclusione, lo sforzo economico, sicuramente di notevoli dimensioni, è stato sostenuto allo scopo di rilanciare una manifestazione di fondamentale importanza per le strategie aziendali della RAI - quale il Festival di Sanremo il successo ottenuto ha confermato la bontà delle scelte effettuate. Quanto alla previsione di un tetto al compenso previsto per chi lavora in RAI, richiesto in una delle interrogazioni, si ritiene di avere in parte già risposto, rilevando la difficoltà per un'azienda presente sul mercato nel sottrarsi alle regole della concorrenza per quanto riguarda i corrispettivi relativi alle prestazioni artistiche. In ogni caso, in termini di principio, si potrebbero mettere allo studio misure tali da estendere anche alla concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico i limiti ipotizzati per le retribuzioni dei dirigenti del settore pubblico. per quanto riguarda la trattativa commerciale relativa alla cessione di alcuni diritti, è da rilevare come questa sia avvenuta parallelamente ma separatamente da quella sul compenso per la partecipazione al Festival, riguardando esclusivamente il segmento *home video* di parte del materiale delle teche della RAI. La RAI, quindi, mantiene intatto e totalmente utilizzabile in perpetuo su ogni piattaforma trasmissiva (analogica, digitale terrestre, digitale satellitare, internet, videofonini, *pay-tv*, radio eccetera) il proprio archivio con le prestazioni di Roberto Benigni, con il quale si è stabilito un rapporto fondamentale e strategico, la cui interruzione costituirebbe un danno in termini economici e di immagine. Su tale problematica, che, come detto, non riguarda il Festival di Sanremo, bensì una operazione commerciale effettuata dalla RAI, sono state chieste alla concessionaria pubblica ulteriori delucidazioni, posto che, a quanto è dato conoscere, l'attuale consiglio scaduto e in carica per la normale attività ordinaria ha deciso di sottoporre la questione al nuovo consiglio che si dovrà insediare per le valutazioni e le eventuali determinazioni di competenza.

Presidente, onorevole Romani, credo che la gente comune dimentichi quasi tutto. In Italia, poi, siamo tutti molto buoni e, quando qualcuno fa sorridere, la gente perdona e comprende. Benigni

Benigni è particolarmente attento anche alla cura dei propri affari. Ci sono allora due questioni che non tornano.

Benigni, in questo caso, ha pagato 453 euro al minuto, che, moltiplicati per i 750 minuti oggetto della questione dei diritti, fanno i circa 340.000-350.000 euro euro pattuiti per quella mezz'oretta di risate elargita a Sanremo. Constato positivamente che c'è un risparmio di 100.000 euro rispetto a quanto speso l'anno prima per la sua partecipazione alla La seconda questione è che la RAI cede normalmente i diritti per le immagini per cinque anni e non in esclusiva, ma Benigni ottiene vent'anni di diritti in esclusiva. Cioè, la RAI non può usare quelle immagini per l'*home

nazionale di inestimabile valore, che acquisisce ulteriore importanza, se consideriamo che può essere - anzi, è stato sicuramente - accumulato negli anni anche grazie al pagamento del canone. Allora, ci domandiamo: chi paga per questo regalo a Benigni? Chi paga per questo pessimo affare commerciale realizzato dalla RAI? Chi paga, il direttore generale Cappon, che ha ignorato più volte l'osservazione dell'amministratore delegato di Rai Trade?

soprattutto) avremo qualche piccolo problema relativamente al contratto in essere sulla cessione dei diritti. Secondo la notizia di agenzia, la direzione di RAI Italia ha comunicato che questa sera la puntata di "Annozero" non potrà essere trasmessa; nella puntata, infatti, vi sarebbero dovuti essere dei filmati di Roberto Benigni di cui non sono stati concessi i diritti di trasmissione internazionale. Dato che lei è un esperto di questioni televisive, forse sarà il caso di rivedere la risposta che gli uffici hanno preparato oppure le indicazioni che le hanno offerto gli uffici della Rai per rispondere in Parlamento. Noi cosa faremo? In Commissione di vigilanza Rai, come capogruppo del PdL, chiederò di verificare tutte le possibilità di rinegoziare quel tipo di contratto, cioè quello stipulato con Roberto Benigni. Ci piacerebbe prendere come esempio quello stipulato con Mina, un mito sicuramente pari a Benigni: ebbene, quel contratto prevedeva diritti non esclusivi per dieci anni con una compartecipazione da parte della RAI al 30 per cento Quindi, riteniamo che occorra moralizzare anche la RAI, partendo proprio dai contratti ad esempio per le produzioni esterne, dai compensi dei conduttori, legandoli ad esempio - ed è questa un'altra proposta che andremo ad avanzare - allo *share* che registra la loro trasmissione oppure all'*appeal* che la trasmissione stessa esercita verso gli investitori pubblicitari. L'ultimo appello che faccio, in scadenza di questi pochi minuti a disposizione, è che mi auguro che i colleghi del centrosinistra possano quantomeno rapidamente

per poter ripartire e mantenere un rapporto internazionale anche con i *broadcasting* europei.

sullo spezzamento dei treni di tipo ETR 500, si deve rappresentare che si è trattato di un intervento automatico del sistema di sicurezza all'avviamento della marcia, avendo il personale di condotta lasciato erroneamente attivo anche il sistema di protezione di coda. Questa condizione, vietata dalle norme d'uso, ha provocato un effetto risonanza, che si è innescato in fase di avvio del convoglio, quando le due locomotive erogano un elevato sforzo di trazione nella stessa direzione, con una contemporanea frenatura rapida automatica dalla locomotiva di coda. In ogni caso, dall'analisi dell'evento emerge chiaro che lo spezzamento si può verificare solo se il treno è fermo e viene avviato con notevole sforzo di trazione. Da questa considerazione si può escludere qualunque connessione con la sicurezza di circolazione. II provvedimento assunto per fronteggiare questa tipologia di errore del personale è stato adottato in data 24 luglio 2008, allo scopo di evitare il ripetersi di situazioni analoghe, ed è stato quello di rendere possibile l'uso di una sola chiave per le due piastre delle locomotive, in modo che possa esserne attivata solo una per volta. Questa disposizione è stata comunicata, come previsto, anche all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Si comunica inoltre che il giudice per le indagini preliminari ha archiviato il procedimento aperto su questi due episodi in quanto l'evento di pericolo non risulta essersi verificato. Da quanto risulta appare quindi che non sono state riscontrate carenze di sorta nel processo manutentivo dei treni ETR 500 in questione e che la sicurezza di viaggiatori e lavoratori non è mai stata a rischio. D'altra parte, in merito al sistema SCMT che realizza una protezione automatica della marcia del treno, si informa che, da quando è iniziata l'installazione di tale sistema sulla rete ferroviaria italiana (2003) e sul materiale rotabile di Trenitalia ivi transitante, gli incidenti interessanti la circolazione ferroviaria si sono ridotti di oltre il 65 per cento, consolidando il primato dell'Italia a livello europeo. Sotto l'aspetto della sicurezza connessa alle condizioni di lavoro dei macchinisti, si premette che in tutto il mondo, pur non disponendo dei sistemi di sicurezza avanzati come quelli installati sulla rete e sui treni di Ferrovie dello Stato, si utilizzano moduli di condotta con un solo macchinista. Si informa che 1'orario di lavoro, secondo 1'attuale normativa contrattuale applicata da Trenitalia, prevede limiti alla condotta dei treni di 7 ore per servizi di andata e ritorno e di 4 ore e 30 minuti per i servizi di sola andata o di solo ritorno. Per quanto di competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito agli episodi di cui trattasi e ad altre problematiche concernenti le porte di accesso delle carrozze e la manutenzione, è intervenuto direttamente, non solo a fronte dei propri compiti

per conseguire la necessaria efficienza ed efficacia dei processi volti al mantenimento di idonei livelli di sicurezza. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ha comunque effettuato immediati accertamenti diretti, finalizzati a verificare la necessità di interventi urgenti. Fatto salvo l'inconveniente tecnico avvenuto, va rilevato che, per entrambi i convogli per i quali si è verificato lo spezzamento, non sono emerse non conformità di attuazione dei programmi manutentivi. In particolare, i "tenditori" vengono revisionati fuori opera anche con sistematici controlli non distruttivi ed eventualmente sostituiti in occasione degli interventi di manutenzione. Per quanto riguarda il più recente episodio di spezzamento avvenuto il 24 gennaio 2009, sebbene non citato nell'interpellanza, si rende noto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha immediatamente attivato apposita indagine nominando una commissione composta da tecnici esperti dell'organismo investigativo istituito presso il Ministero stesso. La commissione di indagine sta procedendo ai primi esami ed accertamenti sul materiale rotabile interessato e sulla specifica documentazione acquisita. L'esame preliminare degli elementi raccolti sembrerebbe poter escludere che la rottura del tenditore fra la 5a e 6a carrozza del treno possa essere avvenuta a seguito dell'azionamento del freno d'emergenza posto a disposizione dei viaggiatori. Ciò in quanto dalle registrazioni risulterebbe che tale dispositivo sia stato attivato circa 15 minuti dopo l'avvenuto spezzamento. Per la valutazione definitiva sulle dinamiche dell'incidente occorrerà attendere la conclusione dell'inchiesta che, presumibilmente, avverrà entro 4-5 mesi. Per quanto riguarda la manutenzione e i controlli ai fini della sicurezza, è previsto, a determinate scadenze, sia in termini di percorrenze che temporali, ed in ottemperanza a quanto stabilito dai progettisti/costruttori del materiale rotabile e a quanto previsto dalle norme di carattere generale, il rientro dei rotabili presso le officine di manutenzione per l'esecuzione delle operazioni previste nei piani di manutenzione. I Piani di manutenzione, che fanno riferimento ai manuali di manutenzione redatti dai progettisti/costruttori del materiale rotabile, sono depositati anche presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF), che, nel merito, dispone delle verifiche sulla conformità delle attività di manutenzione presso le officine di Trenitalia. Nei Piani di manutenzione del materiale rotabile per le attività inerenti la sicurezza, contrassegnate in maniera evidente con la lettera «S», c'è la descrizione delle operazioni, procedure e strumenti necessari per la corretta esecuzione; la tracciabilità dell'avvenuta effettuazione degli interventi è registrata sui documenti aziendali e sul sistema informatico di supporto alla manutenzione. Gli operatori addetti all'esecuzione delle attività in parola, opportunamente formati attraverso periodici corsi di aggiornamento professionale, sono registrati nell'Albo dei manutentori di sicurezza il cui aggiornamento viene periodicamente notificato all'Agenzia nazionale Per quanto concerne la sicurezza della circolazione ferroviaria, è importante cogliere l'occasione offerta dai senatori interpellanti per fornire un quadro di quello che è oggi il ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle diverse autorità presenti nella materia. Preliminarmente, si fa presente che con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è stata istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) a cui sono assegnati i compiti di Autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha funzioni di indirizzo e sorveglianza dell'Agenzia stessa nonché, attraverso apposito organismo investigativo, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti. In attuazione del decreto legislativo istitutivo dell'Agenzia, sono stati emanati e sono in corso di pubblicazione separati regolamenti, che prevedono l'assetto organizzativo e l'adozione dello statuto, nonché l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia. In considerazione di quanto sopra e tenuto conto dell'attuale transizione verso le nuove tecnologie di sicurezza e del conseguente attrezzaggio in corso della rete ferroviaria e dei rotabili con le tecnologie per la sicurezza ed il controllo della marcia dei treni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato un apposito Atto di indirizzo, in base al quale 1'Agenzia ha correttamente avviato le proprie attività e sta quindi rilasciando le certificazioni di sicurezza per la circolazione del materiale rotabile, ed ha assunto importanti decisioni, in particolare circa l'utilizzo di dispositivi atti al controllo della vigilanza del macchinista nell'ambito del sottosistema di bordo dei rotabili. L'Agenzia, inoltre, si è immediatamente adoperata per la soluzione delle principali criticità relative alla sicurezza della circolazione ferroviaria emerse nel corso dell'attività ispettiva avviata, quali, ad esempio, le questioni relative alle porte di accesso delle carrozze adibite al trasporto viaggiatori ed alle operazioni di manutenzione svolte dalle imprese ferroviarie. L'Agenzia, infine, si è attivata per favorire l'attuazione dei programmi delle imprese ferroviarie per il completamento della installazione a bordo dei treni dei sistemi di protezione della marcia del treno. Il Ministero, attraverso la Direzione generale per il trasporto ferroviario, che svolge operativamente le funzioni di vigilanza sull'Agenzia, collabora attivamente alle attività avviate dall'Agenzia stessa. In particolare, poiché la ripartizione delle attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria è di fondamentale importanza per il presidio della sicurezza, presso il Ministero sono stati aperti diversi tavoli di confronto con la partecipazione dell'Agenzia, di RFI SpA, gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, e dei principali operatori del settore (tra cui Trenitalia e ASSOFER, associazione che rappresenta i proprietari di carri ferroviari) in ordine alla manutenzione dei rotabili ed alla ricognizione delle competenze in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia. Nell'ambito delle strutture ministeriali opera l'organismo investigativo preposto allo svolgimento di indagini finalizzate a fornire raccomandazioni per il miglioramento della sicurezza ferroviaria e la prevenzione di incidenti. L'organismo investigativo, le cui funzioni sono previste e disciplinate dal medesimo decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, istitutivo dell'Agenzia, ha prontamente avviato le proprie attività. Al fine di implementare le proprie funzioni e di poter assicurare un pronto intervento del Ministero in caso di incidenti ferroviari, l'organismo investigativo si è dotato di un aggiornato elenco di esperti in grado di assumere il ruolo di investigatore (quindi (quindi indipendenti dai gestori dell'infrastruttura ferroviaria, dalle imprese ferroviarie e dall'Agenzia), reperiti non solo presso le strutture centrali e periferiche del Ministero, ma anche presso università, genio ferrovieri e altri organismi operanti nel campo. In ottemperanza a quanto previsto dalle norme comunitarie, l'organismo partecipa ai gruppi di lavoro in materia presso l'Agenzia ferroviaria europea, ha stabilito i criteri per l'avvio di un'indagine in caso di incidenti ed inconvenienti ferroviari, ed ha aperto appositi tavoli di confronto con gli operatori, anche al fine di regolare i necessari flussi informativi. L'organismo investigativo, nel corso del corrente anno, oltre ad aver attivato indagini su specifici incidenti ed inconvenienti di rilievo, ha avviato una apposita indagine di carattere più generale in ordine al fenomeno degli svii, ossia i deragliamenti. Da ultimo, si evidenzia che Trenitalia ha già attuato alcune azioni correttive, mentre l'Agenzia ha già condotto un primo esame della questione sulla base degli elementi disponibili, impartendo alcune ulteriori indicazioni a Trenitalia, fra cui quella di estendere i provvedimenti ad altre tipologie di treni analoghe agli ETR 500.

quindi, da capire perché questo treno si sia spezzato in due parti. Poiché abbiamo un comunicato delle Ferrovie dello Stato che parla di atto doloso,

fu lo stesso ingegner Moretti a dichiarare, in una nota ufficiale, che probabilmente vi erano dei difetti costruttivi di minore

al riparto della somma in base ai contratti di servizio che le Regioni avrebbero stipulato con lo

II decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 25, comma 2, stanzia 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 «per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario». La ripartizione di tali fondi è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Peraltro, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, come modificato con legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, all'articolo 27 ha disposto che tali risorse siano interamente destinate alla finalità sopra indicata, sancendo che i contributi all'acquisto del materiale rotabile per il trasporto regionale - che con la legge n. 2 del 2009 erano stati previsti a valere sulle risorse in questione siano attribuiti a valere sui fondi di cui al comma 1 dello stesso articolo 25 (fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie Lo scorso 17 dicembre, a valle dell'emanazione del decreto-legge n. 185, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha tenuto un incontro con le Regioni

si è determinato di attribuire interamente i 480 milioni di euro ai servizi regionali, in misura di 430 milioni alle Regioni a Statuto ordinario e 50 milioni a quelle a Statuto speciale. Il successivo 18 dicembre, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha elaborato un documento, presentato alla Conferenza unificata che si è tenuta in pari data e che ratifica la ripartizione di cui sopra. Va osservato che nel documento della Conferenza delle Regioni è specificato che: «la ripartizione dei 430 milioni di euro tra le singole Regioni sarà in proporzione ai trasferimenti storici, in considerazione del fatto che le risorse da ripartire sono finalizzate a garantire l'attuale livello dei servizi». Si può dunque concludere che le Regioni, nel loro complesso, concordino sulle esposte modalità di ripartizione dei fondi in parola, che anzi riflettono pienamente la proposta da esse formulate. Il successivo 12 gennaio, per quanto di competenza di questo Ministero, è stato trasmesso al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze uno schema di decreto di ripartizione, i cui contenuti sono diretta funzione di quanto sopra evidenziato.

Ringrazio il Sottosegretario per le informazioni che mi ha dato. Evidentemente i miei appetiti sono maggiori di chi governa di chi governa nella mia Regione: credo che chiedere di più da parte di chi ha di meno sia normale e molto civile.

che questo è quanto è stato chiesto. Cosa devo rispondere, Sottosegretario? Ho capito che non posso che rispondere questo. Se fossi stato io a capo di quella Regione, avrei tentato di ottenere qualcosa di più, perché mi sembra che